Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori,

non riesce a dirimere con definizioni chiare e precise. Mai più emergenza, mai più dubbi atroci e laceranti: per noi la vita è intangibile, indisponibile e va assistita come il bene più prezioso. Il nostro primo diritto di libertà è quello di nascere e di vivere e pertanto è un diritto da difendere fino al momento estremo. Vi può essere forse un limite, ove il valore della vita in qualche modo decade? Non credo che esista un momento nel quale un aggettivo sia sufficiente a diminuire il dato fondamentale del sostantivo del vivere, dell'essere e del partecipare non vi è un momento compassionevole che possa in qualche modo attutire il valore intrinseco della vita medesima. Gli aggettivi non possono eliminare questo dato. Allora, la risposta che diamo è no, perché la vita va difesa, conservata ed assistita. Certamente vanno modificati i contesti nei quali le difficoltà si determinano. Anche i colleghi dell'opposizione ieri sono intervenuti dimostrando questa sensibilità e questo tipo di attenzione.

quando abbiamo ritenuto che qualunque mezzo in grado di alleviare il dolore potesse offrire nelle situazioni terminali, estreme o importanti un aiuto tecnologico e scientifico affinché il dolore non mortificasse il quotidiano

dolore? Su questo tema dobbiamo appassionarci. Qualsiasi mezzo, qualsiasi momento e qualsiasi occasione organizzativa, tecnologica ed innovativa, se portano un contributo

eminenti costituzionalisti ci hanno ricordato che si tratta di un momento fondamentale che deve essere consegnato alla disponibilità di ognuno affinché possa vivere nella maggiore dignità possibile fino all'ultimo momento della propria vita. Scelga questo Parlamento per noi, in modo semplice, senza tante altre parole e che, così come si dice nella premessa della mozione, non si muoia mai per fame e per sete in questo Paese.

che si conferma anche nella scienza e nei nuovi mezzi e che va oltre: l'*homo faber* diventa *homo sapiens* e trasforma - ripeto - la tecnologia come momento arricchente per migliorare fino all'ultimo la qualità della vita.

non sfugga a nessuno la complessità del momento nonché le grandi sfide che che abbiamo davanti, in un mondo dove culture diverse si stanno confrontando per trovare un modello di convivenza globale, all'interno di un fortissimo processo di trasformazione. Questo processo di confronto e di ricerca richiede fatica, richiede anche momenti di crisi rispetto alle idee e alle credenze; esige grande coraggio nel giocare fino in fondo dentro la società e dentro le trasformazioni e i valori in cui crediamo. Del resto, sappiamo che questa è una società che ha bisogno di valori e non di dividersi, ha bisogno di ritrovare una nuova condivisione e un solido orizzonte valoriale in cui riconoscersi tutta. tutta. Se manca un'idea di bene comune, che è da costruire, le società tendono a secolarizzarsi ulteriormente, si frammentano, involvono, diventa più conflittuale, più secolare; non trova più la forza del suo riscatto e Dio sa quanto in questo momento le nostre società, di fronte alle crisi che abbiamo di fronte, hanno bisogno di trovare energie e forza per unirsi, per riscattarsi e ripartire. Servono quindi valori condivisi da proporre a questa nostra società confusa ed è necessario che questi valori vengano testimoniati da noi con coerenza, cari colleghi della Lega, del Popolo della Libertà, noi tutti.

La vita umana è uguale tutti giorni e, se consideriamo questo come un valore fondante della nostra società dall'inizio alla fine, questo dobbiamo testimoniare. La vita umana non può essere piegata a strumentalizzazioni ideologiche. Questo deve essere chiaro anche nel momento in cui affrontiamo il tema del testamento biologico, così come quando abbiamo affrontato altri temi "faticosi", come quello della sicurezza, nei giorni scorsi. Ecco perché in questo momento sia i credenti che i non credenti sono chiamati a portare dentro questo disegno di legge il loro contributo più vero. È chiaro che dobbiamo cercare di trovare anche su questi temi etici, che interessano tutta la società, una capacità di sintesi alta, piuttosto che portare avanti battaglie radicali, che rischiano di dividere noi e la società e che, alla fine, non risolvono in fondo i problemi della nostra società. *(Applausi del senatore Astore).* Se radicalizziamo i problemi faremo una legge buona per alcuni e cattiva per altri. Noi, nel limite del possibile, testimoniando il valore della vita, dobbiamo varare una legge buona per la maggior parte dei nostri cittadini. La debolezza sta nel dividere la società; la forza sta nel tentare di tenerla unita, oggi come oggi, in questo momento di crisi. E solo due culture molto forti, con quella cattolica e quella liberale, possono scontrarsi, ma poi incontrarsi in una condivisione e cercare insieme orizzonti condivisi di valori, senza la paura di cedere nemmeno un centimetro della propria identità, ma con la certezza di avere almeno tentato di giovare al progresso della nostra società. Ecco perché il concetto di autodeterminazione, ad esempio, caro alla cultura liberale,

L'idea che comunque il concetto di una società solidale debba confrontarsi con quello di una società liberale è un qualcosa che dobbiamo affrontare all'interno di questo Parlamento se vogliamo trovare soluzioni condivise non solo sui temi etici, ma anche su quelli della rinascita economica e sociale del nostro Paese. Ed ecco perché anche su temi delicati come quelli a sfondo etico dobbiamo provarci, cari colleghi, dobbiamo provarci tutti. Abbiamo un dovere morale e questo è lo spirito della nostra mozione. Con questo spirito ci presentiamo al Parlamento. Si tratta di una mozione faticosa, che cerca davvero di tenere insieme queste due grandi culture, queste due grandi tradizioni, l'orizzonte di un bene comune verso il quale vogliamo andare. Sono d'accordo con tante cose dette dal senatore Saccomanno. Chi di noi non è a favore della dignità della vita, fino in fondo, e

fino in fondo, quindi aumentare la rete degli *hospice,* potenziare le cure palliative; non dobbiamo prenderci in carico il malato solo con i disegni di legge, ma nella società di tutti i giorni, nella nostra quotidianità. Bisogna anche investire risorse per fare tutto questo

consideriamo come un principio di precauzione il fatto che vi sia un'alleanza terapeutica fra medico e fiduciario; prevediamo l'obbligatorietà del fiduciario; prevediamo una scadenza precisa per la DAT, che dev'essere di cinque anni; prevediamo anche - e questo è un principio fondamentale su cui tentiamo di fare una sintesi - che, senatore Saccomanno, idratazione e nutrizione siano garantite al paziente come sostegno vitale, non come trattamento sanitario, fino alla fine della vita. vita. Si tratta di un passaggio culturale fondamentale, ma altresì non possiamo negare, in ossequio al principio di autodeterminazione, che ci possa essere qualche cittadino che, dichiarandolo in modo esplicito,

e quindi alla redazione di un testo normativo che sia veramente di sintesi delle varie sensibilità che rappresentano il nostro Paese, devo svolgere alcune considerazioni e le svolgo, signor Presidente, da cittadino di uno Stato laico, da cattolico credente, da medico, da parlamentare. Le svolgo con un senso di tristezza per le modalità con cui si è giunti alla discussione di un tema così delicato e complesso, con il rispetto per chi si sente di avere certezze e anche con il travaglio di chi, come me, come noi, non pensa di darle.

quanto abbiano pesato in questa sconcertante vicenda le questioni di principio e quanto le strumentalizzazioni di parte, volte spesso a fini diversi da quelli dichiarati. Sono temi sui quali non servono esasperazioni ideologiche, scontri fra opposte fazioni, sovraesposizione mediatica di vicende singole. La responsabilità di dividere il Paese di qua i difensori della vita e di la i fautori della morte - è quanto di più pericoloso si poteva immaginare che accadesse e purtroppo è quello che sta accadendo oggi in quest'Aula del Senato. Il Paese aveva bisogno di altro: aveva bisogno di un atto di laicità, di un segnale forte dell'autonomia dello Stato di diritto nel deliberare il difficile equilibrio tra scienza e individuo. Nessuno vuole disconoscere, come è stato richiamato dai banchi della maggioranza, la centralità della morale nella vita degli uomini, del confine tra la vita e la morte, del sacro, del diritto. Al contrario, si vuole riconoscere questa centralità e riaffermarla nel pluralismo delle convinzioni, delle idee, delle religioni, delle visioni del mondo che una convivenza civile alla base di uno Stato di diritto deve saper mediare, regolare, ma soprattutto garantire e proteggere. Questa è materia sulla quale i legislatori di un Paese normale dovrebbero fare lo sforzo di maturare le proprie decisioni in un clima il più possibile di confronto pacato, sapendo ognuno di noi che non c'è una soluzione esclusiva e indiscutibile, ma solo una difficile ricerca, in una società pluralista, di decisioni il più possibile condivise. Nella legalità costituzionale, dove sono in discussione contemporaneamente i poteri di uno Stato di diritto e i diritti individuali e fondamentali delle persone, il Parlamento non può ignorare l'intangibilità dei provvedimenti giudiziari definitivi. I giudici con alcune decisioni, in particolare con la sentenza cardine della Corte di cassazione, hanno potuto ricostruire quegli elementi che già consentono di arrivare ad un principio giuridico definito, cioè il diritto di rifiutare le cure e di morire con dignità, che è cosa ben diversa dal diritto alla morte o dalla deriva eutanasica dei nostri valori. La dignità è quella di chi deve essere rispettato nelle sue decisioni e nel suo essere persona e non di chi deve vedere la propria sopravvivenza nelle fasi finali resa obbligatoria da un'imposizione di Stato. La dignità è che la scienza e l'etica collettiva non devono mai rischiare di sostituirsi alla persona, di farne una cosa, un oggetto di trattamenti senza speranza o destinataria di imposizioni. La scienza e la tecnologia medica hanno compiuto progressi che hanno stravolto il morire, essendo diventate per certi aspetti le vere proprietarie della definizione di questo confine. Nei decenni passati non c'era bisogno - né ci sarebbe stato - di fissare limiti all'accanimento terapeutico, all'alimentazione artificiale parenterale di pazienti che in stato vegetativo permanente non percepiscono più la sete e la fame. Non c'era la distinzione enorme tra l'individuo cosciente, che può invocare la libertà di cura prevista dalla nostra Costituzione, e chi chiede il rispetto di questo diritto anche quando non vi è più coscienza, chi chiede il permanere di un diritto prima della morte biologica. Perché di questo si tratta. Vi è poi il merito della questione legislativa. Mi rivolgo ai colleghi della maggioranza che hanno così tante certezze: ma davvero noi pensiamo che una norma rigida e assoluta come quella di cui si sta discutendo e che è contenuta nella mozione di maggioranza, che imporrebbe in ogni caso e in qualunque circostanza il divieto di interrompere idratazione e alimentazione parenterale delle persone in stato di fine di vita, sia la soluzione più giusta? O non sarebbe meglio lasciare degli spazi anche a valutazioni di scienza, di coscienza, adeguate ai casi concreti che sono sempre diversi tra di loro? Su questo punto la Costituzione pone alcuni limiti invalicabili. L'articolo 32, sancendo il diritto alla salute e il principio per cui nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge (e la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana), fa conseguire che anche l'alimentazione e l'idratazione artificiali non possono essere forzate, cioè imposte contro la volontà della persona interessata. Sono in gioco valutazioni di estrema delicatezza, in cui la scienza e la coscienza dei medici e la coscienza dei familiari della persona interessata non possono essere sottoposte a nessun imperativo di Stato. Prima di noi altri Paesi hanno adottato il testamento biologico (Francia, Spagna, Svizzera, Olanda, Belgio, due Stati del Canada), mentre le direttive anticipate hanno valore legale in alcuni Stati dell'Australia e degli Stati Uniti d'America. In Inghilterra e in Germania, pur non essendoci una specifica normativa al riguardo, il testamento biologico trova attuazione nella pratica e conferma nella giurisprudenza.

quale ha ricordato che, se una cura non porta alcun beneficio, può essere legittimamente interrotta; che in uno stato vegetativo permanente l'alimentazione e l'idratazione artificiali sono assimilabili a trattamenti medici; che, quindi, non è giustificabile, secondo qualunque principio etico e religioso, l'accanimento contro un povero corpo martoriato, tenuto artificialmente in un limbo. Vedete, colleghi, caro Presidente: la fede cristiana sa dare anche delle profonde lezioni di misericordia e di pietà cristiana. Signor Presidente, nel presentare la mozione n. 88, il Gruppo dell'Italia dei Valori ribadisce che è necessaria una legge sul testamento biologico, ma crediamo che soltanto in una prospettiva laica, rispettosa delle diversità, dubbiosa senza ipocrisie, soltanto in questa visione, una legge del genere potrà essere un progresso e non invece un'occasione di lacerazioni per un Paese che ha bisogno, oggi più di prima, di unità morale.

In questo momento il testo si legge in tale maniera: «impegna il Governo a garantire che, in attesa dell'approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di fine vita, l'alimentazione e l'idratazione...»; chiedo

in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere negate da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

Grazie,

perché ritengo la vita un dono di Dio e che solo Dio è l'arbitro unico della nostra vita. Dunque, mi è molto facile, non mi nascondo dietro considerazioni ambigue. Come politico, invece, penso che abbiamo una società così organizzata che forse potevamo fare di più. La nostra società ha teste di cuoio, pronte ad intervenire in molti casi.

Abbiamo i «Medici senza frontiere», che però non sono riusciti ad arrivare a portare un bicchiere d'acqua ad Eluana. Ecco, queste cose mi hanno sconcertato, mi rendono mi rendono triste, nel mondo della politica in cui vivo, e non posso far altro che ripetere le parole di un vescovo che dice: «Dio accolga e perdoni chi l'ha portata a questo punto». E di questo perdono penso che abbiamo bisogno tutti, sia quelli che stanno seduti a destra sia quelli che stanno seduti a sinistra in Parlamento, perché assieme forse non abbiamo fatto abbastanza per questa ragazza.

Ciò impone pacatezza nei toni ed equilibrio dei giudizi. C'era un aspetto giuridico una sentenza e, in uno Stato di diritto, i pronunciamenti dell'ordine giudiziario al loro ultimo grado devono essere rispettati.

Permettetemi di dire che ho assistito al dramma di Eluana e di Beppino Englaro con la sensibilità di chi è loro concittadino, sono stato sindaco di Lecco per nove anni. Ho visto bene come la comunità lecchese ha vissuto questi momenti, tra contrasti e lacerazioni e ho ragione di credere la buona fede ispiri all'uno e all'altro schieramento, se così si possono definire, un diverso atteggiamento della coscienza. Ma c'è anche da dire che il fatto di specie è stato assolutamente inconsueto, perché non si trattava di schierarsi pro o contro l'accanimento terapeutico, bensì di procurare la fine di una vita, sospendendo cibo e acqua. In un Parlamento composto da uomini liberi, ci apprestiamo a legiferare non intorno ad un caso, anche se quel caso dolorosissimo ci aveva messo fretta;

quello di Eluana rimanga l'ultimo caso di morte per sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione. Non tocca a noi indagare ulteriormente su quella che era stata la volontà di Eluana messa in discussione in questi giorni; ma è certo che il cammino compiuto a Udine, nonostante il sostegno del diritto, aveva più il carattere della morte che della vita. La forza del diritto può essere fragile se asseconda un disegno che apre orizzonti inquieti e crea pericolosi precedenti. Il ragionamento intorno alla vita deve prendere spinta dalla considerazione che essa è un bene inestimabile e inalienabile e sulla quale non c'è arbitrio umano, specie per chi è cattolico credente. Spero che la nuova legge che il Parlamento approverà porrà soluzione ad un *vulnus* legislativo. Spero anche che sia una buona legge nella convinzione che vi sia affermato il primato della vita, che deve essere l'obiettivo e la *ratio* di questo nostro provvedimento. Mi sento altresì di dire, in conclusione, che la contrapposizione che sta vivendo e che sta coinvolgendo l'intero popolo non dovrebbe impedire che ciascuna opinione abbia cittadinanza in uno Stato laico, che laicamente chiama il Parlamento sovrano a pronunciarsi su una questione di coscienza, non su un caso, ma su una condizione fragile dell'uomo che non possiamo lasciare in balìa di opinioni, di stati d'animo o di sentimenti.

vorrei distinguere, nel mio intervento, la parte che svolgo nella mia veste di politico e quella che svolgo come credente. Non perché questo mi conduca a due conclusioni diverse, ma perché mi sembra necessario sottolineare una distinzione tra i due piani del discorso, che troppo sovente è ignorata o trascurata. Nella veste di membro laico di un Parlamento laico ritengo che la legge debba limitarsi a definire il confine al di qua del quale c'è sicuramente vita umana da difendere con ogni mezzo, e il diverso confine al di là del quale il corpo umano può e deve essere considerato a tutti gli effetti morto. Questi sono i soli *certi* *fines*, i confini sicuri, che un ordinamento civile moderno può e deve porre. Ed essi non sempre coincidono tra loro. Dico che non coincidono sempre perché tra di essi vi è talvolta una sorta di zona grigia, una zona di ragionevole opinabilità (quella che gli anglosassoni chiamano *band of reasonableness* delle opzioni possibili), dove possono verificarsi una infinità di situazioni-limite particolari, la cui qualificazione è controvertibile. In questa zona, a ogni cittadino deve essere consentito, con l'assistenza del medico o di altro consigliere di sua scelta, agire secondo la propria coscienza. Detto questo, e parlo ancora come membro laico del Parlamento di una Repubblica laica, rispetto e difendo il diritto di chiunque, nel nostro Paese, quindi anche dei vescovi e in generale del magistero ecclesiastico cattolico, come ovviamente degli esponenti di qualsiasi altra chiesa o comunità religiosa, di esprimere liberamente la propria opinione sul discrimine tra vita e morte, tra vita biologica e vita umana, o persino su che cosa la legge dovrebbe stabilire al riguardo fin nel dettaglio: dissento recisamente da chi vede sul piano istituzionale, dal punto di vista laico, da cui sto parlando, parlando, negli interventi delle autorità religiose su questo terreno un'ingerenza indebita o comunque una scorrettezza. È come cristiano (forse sarebbe meglio dire come persona impegnata a coltivare intensamente il patrimonio plurimillenario della tradizione biblica), è in questa veste che mi rammarico di interventi del tipo di quelli che la chiesa cattolica con frequenza compie su ciò che questo Parlamento deve o non deve fare. Ed è in questa veste che mi rammarico di un Governo che a questi interventi assoggetta programmaticamente e sistematicamente il proprio agire; incurante, oltretutto, del fatto che della nostra tradizione biblica non è depositaria soltanto la chiesa cattolica, ma anche altre, come quelle protestanti e in particolare quella valdese; ne è depositaria pure, e da molto prima, la comunità ebraica. E tutte queste dalle Scritture traggono insegnamenti di etica politica talora profondamente diversi rispetto alla chiesa cattolica. In consonanza con tanta parte di questa grande comunità di persone che nella tradizione biblica cercano il senso della propria vita, penso che la testimonianza di una chiesa cristiana non debba mai consistere nell'indicare la soluzione giuridico-legislativa specifica da preferire, né tanto meno le concrete modalità dell'impegno politico; penso che essa invece debba educare i cristiani all'esercizio responsabile della loro coscienza, lasciando che proprio quest'ultima, la coscienza, resti il punto di riferimento fondamentale per ciascuno di loro nelle scelte politiche, giuridiche, tecniche e professionali. Pietro Scoppola amava citare, a questo proposito, un'affermazione del Concilio Lateranense IV del 1215: «*Quidquid fit contra conscientiam aedificat ad Gehennam*»" (qualsiasi cosa che si faccia contro la propria coscienza prepara all'inferno), concetto ultimamente ribadito dalla *Gaudium et Spes* del Concilio Vaticano II. Nelle materie che, secondo il Vangelo, vanno «rese a Cesare» - e tra queste vi è certamente la materia della legislazione civile le scelte operative devono esprimere i valori in cui crediamo attraverso la mediazione della coscienza di ciascuno di noi. «Rendere a Cesare quel che è di Cesare» significa rispettare la laicità dello Stato, della sua politica, della sua legislazione. Questa laicità è sostanzialmente il metodo che consente a tutte le persone di buona volontà di trovare un terreno comune sul quale mettere in comunicazione le loro coscienze, ispirate a fedi e filosofie anche molto diverse tra loro, per cooperare nella ricerca delle soluzioni tecniche, politiche, legislative migliori per il bene del Paese. Quel terreno comune viene meno se c'è qualcuno che su di esso, cioè in quello spazio che il Vangelo ci invita a «rendere a Cesare»,

Con gli occhi di chi legge la Bibbia, vedo in questa pretesa una violazione del secondo comandamento: «Non nominare il nome di Dio invano». Per concludere, chiedo alla Chiesa di affermare con forza il valore della vita, ma di rendere alla scienza ciò che le è proprio. cioè, ai neurologi la valutazione tecnica circa l'irreversibilità della scomparsa di una componente essenziale della vita umana: l'attività cerebrale, la coscienza; lasciare, più in generale, ai medici la scelta del modo concretamente più umano, misericordioso, caritatevole di trattare, nella loro infinita varietà, i casi in cui si determina questa scomparsa irreversibile. È certo compito della Chiesa continuare a educare con rigore e passione le persone ai valori evangelici, ma essa deve lasciare loro - e in particolare a a quelle che sono impegnate negli organi legislativi e amministrativi dello Stato - la libertà di compiere secondo coscienza le scelte proprie della funzione civile o professionale che esse svolgono, confrontandosi in proposito con le persone di fede diversa senza la pretesa di possedere in quel campo una verità rivelata, direttamente attinta dalla volontà divina. Anzi, credo che la Chiesa debba vegliare a che nessuno avanzi questa pretesa, nessuno violi il secondo Comandamento. Al Governo e al Parlamento, invece, chiedo di riconoscere e proteggere, come impone la Costituzione, nella zona tra i due confini due confini (della certezza della vita umana, da una parte, della certezza di morte, dall'altra), quella *band of reasonableness* delle opzioni possibili all'interno della quale ogni cittadino, cristiano o no, deve poter decidere e agire secondo la propria coscienza.

Voglio ringraziare anche, lo dico a nome dei senatori del mio Gruppo, tutti i colleghi del Popolo della Libertà, perché ieri abbiamo dimostrato che su questi temi e su questi valori nella

da questa vicenda con le idee un po' più chiare, nel senso che non si può andare avanti con le strumentalizzazioni; non è giusto né corretto arrivare agli scontri politici quando si parla di queste cose.

- e scusate se lo dico anche ai colleghi del centrosinistra che erano contrari ad approvare questo provvedimento - perché un Paese civile non può permettere che avvengano simili cose, quando

a tutte le nostre famiglie e alle comunità, le quali, anche loro, stanno dibattendo su questi argomenti. Non possiamo noi accendere la miccia, dobbiamo invece cercare di usare l'intelligenza e il buonsenso

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, voglio provare a recuperare la necessaria serenità di giudizio e pacatezza di toni, evitando così di cedere alla facile tentazione della polemica. Voglio anche aggiungere che ho sincero rispetto per le posizioni, pur diverse dalle mie, che in buona fede sono state espresse su questa vicenda. In questi giorni però mi è martellata in testa continuamente una domanda che pongo a voi, colleghi, che non avete condiviso la proposta di una legge che vietasse di togliere il nutrimento e l'acqua a qualsiasi essere umano. Mi rivolgo ovviamente a coloro che non si sono trincerati dietro la motivazione dell'incostituzionalità del provvedimento, ma a coloro che hanno rivendicato la legittimità morale della scelta consentita dalla Corte di cassazione e cioè il porre fine, con l'interruzione dell'alimentazione, alla vita di un invalido grave incapace di intendere e di volere sulla base della richiesta di un genitore. La domanda che pongo a voi è: dove si fissa l'asticella? Se il criterio non è quello del rispetto della persona umana sempre e comunque, perché essa ha un valore superiore non disponibile, quale deve essere il criterio e chi lo fissa? Se il criterio è quello della qualità della vita, sarà sempre discutibile e l'asticella potrà essere abbassata sempre di più. *(Applausi della senatrice Bianconi)*. Allora perché non porre termine anche alla vita degli ammalati di Alzheimer allo stadio avanzato, perché non alla vita di quei vecchi ormai incapaci di provvedere a se stessi? E ancora, perché non abortire un feto gravemente malformato anche al quarto o magari al quinto mese e perché non alla nascita? O magari perché non eliminare uno psicotico grave ed irrecuperabile? O perché non eliminare un condannato all'ergastolo per reati disumani? Sullo sfondo vedo certamente la legittimazione dell'eutanasia e del libero aborto, ben al di là della lettera della legge n. 194 del 1978. L'idea che si legittima è che noi, a certe condizioni, possiamo disporre della vita umana. Ma chi stabilisce quali siano le condizioni? Quando ci si avvia su una certa strada il rischio è che non ci sia più alcun limite al nostro cammino. E se il discrimine sarà il consenso (peraltro qua del tutto inesistente), perché allora non depenalizzare l'aiuto al suicidio, chi abbia fornito assistenza a un uomo che abbia chiesto di essere aiutato a morire? E non vorrei che qualcuno finisca magari un giorno con il tirare in ballo i costi per la società. Ci sarà sempre un economista che proporrà come criterio il rapporto costi sociali e benefici individuali. Questa preoccupazione l'ho già sentita avanzare. Temo che i vostri sforzi saranno vani nel cercare di definire dei limiti, perché sarà facile trovare degli argomenti più efficaci dei vostri per dimostrare che quei limiti sono discutibili e fallaci. Comprendo la filosofia e i valori che ispirano certe logiche; dietro sta un razionalismo illuminista che non crede che l'uomo abbia una dimensione superiore a quella di un semplice aggregato di carne, ossa e sangue. Ma, com'è stato detto, se non riconosciamo in ogni persona l'esistenza di quella dimensione superiore che non dipende dal nostro arbitrio definire o limitare, cede anche l'argine per giustificare la condanna delle peggiori aberrazioni. Di quanto quel confine possa essere facilmente oltrepassato la storia ha già dato tragiche testimonianze. Il rischio è che si apra una voragine in cui finisca con l'essere travolta la nostra civiltà. Allora credo che sia meglio fermarsi e riconoscere che la vita non si può toccare.

la nutrizione e l'idratazione artificiale sono trattamenti sanitari attuati attraverso una sonda gastrica e un intervento chirurgico tipo PEG che necessitano del consenso informato da parte del paziente. Il secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione sancisce la libertà di cura: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessuno caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Io avrei voluto che questi due concetti chiari fossero impegnativi per un Governo e per un Parlamento, per qualsiasi Governo e per qualsiasi Parlamento, affinché appunto venissero seguiti e rispettati i princìpi dell'autodeterminazione e della libertà di cura, nel rispetto proprio del dettato costituzionale, per qualsiasi atto, per qualsiasi provvedimento e per qualsiasi legge

Parlamento, a questo Senato, rispetto ad un salto nel vuoto che rischiavamo di far fare alle istituzioni con l'approvazione di una legge inutilizzabile, scritta male e in fretta, imposta nei modi e nei dal Governo al Parlamento. Ieri sera ci siamo fermati ma oggi, comunque, le emozioni scorrono ancora forti. Sapere che, finalmente, Beppino Englaro è riuscito a piangere a piangere una figlia che ha accompagnato alla sua fine, alla fine che la natura le ha destinato, dovrebbe spingere a usare i toni della ragione. Un appello alla ragione dovrebbe essere quello che, mi auguro, facciamo tutti. Come diceva Goya, il sonno della ragione genera mostri e il rischio, appunto, è quello di produrre non una buona legge ma una legge mostruosa. Il diritto alla vita, più volte enunciato, non può

come sta scritto nella mozione del Partito Democratico, non può divenire un obbligo di cura. Garantire l'alimentazione e l'idratazione: questo deve essere il compito dello Stato e delle leggi e non obbligare a delle cure. Noi saremo chiamati a legiferare su questi temi, su questi argomenti, e mi auguro che la posizione lo farei" non si trasformi in una norma in cui si scriva "tu non lo devi fare, tu non lo puoi fare".

di legge per disciplinare, per regolamentare, per legalizzare quello che oggi è un fenomeno clandestino e illegale, che si verifica nell'Italia che dice di no ma che, invece, si ritrova con persone che muoiono, che

è un concetto più volte ribadito, ma è un concetto che viene stravolto. Infatti, se quella vita umana è indisponibile per l'uomo per chi allora è disponibile? Per lo Stato? Per lo Stato? È disponibile al Governo? Allora quel corpo, che non è disponibile all'uomo, diventa un corpo gestito, disposto, organizzato, nutrito, riempito, svuotato dalle mani dello Stato? appunto - corpi che non sono più individui in grado di scegliere su se stessi, ma corpi in gestione al Governo. Una volta esistevano gli schiavi e i liberi; poi sono scomparsi gli schiavi; oggi ad essersi dileguati sono i liberi. Chissà che faranno ora quelli che nella maggioranza del Popolo della Libertà dicono di essere liberi! *(PD)*. Signor Presidente, io parlo da credente, credente nello Stato di diritto, che è l'unico che può consentire il diritto alla vita

Come molti, magari anche dei presenti, avrebbe potuto, avvalendosi della complicità di un medico, di un avvocato o di un istituto privato, porre fine a quella sofferenza al secondo anno di coma della figlia ed, invece, ha scelto altrimenti: ha scelto di farsi paladino del rispetto delle volontà attraverso l'affermazione della legge, attraverso l'affermazione dell'unica cosa che può garantire a chiunque, comunque la pensi, di potere esprimere il proprio pensiero e farlo diventare una decisione vincolante relativamente alla qualità e alla dignità

a portare a termine entro il 2008 il percorso legislativo relativamente al testamento biologico. Oggi il calendario segna il 10 febbraio e, quindi, ancora una volta si è data ampia dimostrazione del fatto che forse il problema non è quello. Si è piuttosto strumentalizzata ed utilizzata lanciata l'accusa di aver provocato la morte di qualcuno, salvo poi stamani, in esordio di tutti gli interventi, auspicare che si abbassino i toni. Il mio tono è abbastanza basso,

giudaico-cristiani, liberali, ebraici o pienamente musulmani. Questi valori sono sicuramente importanti

ieri, ma almeno 60 anni fa con la nostra Costituzione e, ulteriormente, con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e, ancora, 40 anni fa con il Patto internazionale sui diritti civili e politici o il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, strumenti Quindi, sicuramente sì ai valori umani, ma altrettanto sicuramente sì ai diritti umani. I diritti umani sono universali e l'Italia credo abbia più volte dimostrato a livello mondiale di essere paladina del rispetto di tali diritti, primo tra tutti il diritto alla vita, anche del peggiore delinquente genocidario, sia perché è riuscita in poco tempo a fare adottare lo Statuto del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, che anche per il genocidio non prevede la pena di morte, sia perché due anni fa ha proposto - ed è riuscita a portare a casa con voto straordinariamente ampio in Assemblea generale - una mozione per la moratoria della pena di morte. Stiamo parlando di diritti umani che erano già stati riconosciuti nell'articolo 2 della nostra Costituzione repubblicana, che voglio ricordare, visto e considerato che qui la pratica della legalità costituzionale purtroppo - e questo appartiene tanto alla maggioranza quanto alla minoranza - non alberga nei cuori e nelle menti di molti di noi. qualcuno ha memoria di ciò che è avvenuto questa estate e degli interventi che i radicali hanno svolto in quest'Aula, la denuncia della violazione della legalità costituzionale era, purtroppo, argomento quotidiano in merito alla vicenda della costituzione della Commissione di vigilanza RAI. L'articolo 2 della nostra Costituzione recita: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Ebbene, tra i diritti inviolabili dell'uomo, c'è anche quello di poter

e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno» - ripeto nessuno - «può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. - sottolineo, in nessun caso - «violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana», come codificati nell'articolo 2. È stato detto che c'è chi vuole radicalizzare lo scontro: i radicali non vogliono farlo in alcun modo; si chiamano radicali perché vogliono andare alla radice del problema. Qui il problema non è biologico, il problema è di mantenere intatta la possibilità per il cittadino italiano o per l'individuo che si trovi in Italia di disporre del proprio diritto alla vita e quindi decidere come viverla e fino a quando viverla. Se avessimo avuto la possibilità di andare avanti con il dibattito di ieri sera, emendamento per emendamento, questo sarebbe emerso. Oggi ci troviamo ad affrontare un dibattito ampiamente e profondamente politico, un dibattito che credo dobbiamo a a Beppino Englaro, al quale vanno le nostre condoglianze e i nostri auguri perché il suo esempio ci ha dato forza e quando gli italiani ne sono stati raggiunti credo abbia sollevato in tutti loro un dubbio

ho chiesto per pochi attimi di prendere la parola non per riaprire - non mi compete - un dibattito politico che ieri è stato più che sufficiente, né per parlare nuovamente in modo specifico della povera protagonista di questa vicenda. Eluana ormai, al di là delle nostre parole, si trova dove si trovano le risposte eterne ai quesiti che accompagnano e talvolta angosciano gli anni della nostra vita terrena. Voglio semplicemente aggiungere non nella strada, non in casa, non nella Chiesa, ma nel Parlamento della Repubblica italiana, una parola di ammirazione e di gratitudine profonda non ai soggetti istituzionali o privati a cui ho sentito con il turibolo innalzare incensi in questi due giorni, ma a persone molto più umili e modeste, a quelle suore misericordine che non hanno sposato tesi, non hanno fatto veglie, non hanno partecipato a cortei, non hanno aderito a filosofie, ma nel loro silenzio hanno detto una cosa sola:

non le carte costituzionali, pure importantissime, non i documenti del Parlamento, né le più alte (rispettate o meno) autorità di questa o quella istituzione, ma una o più persone che dicano: ti lascino a me, mi prendo cura io di te. Vada a queste donne silenziose, inimitabili, la parola di una parte, di uno solo, dei membri del Parlamento. E se questa, onorevoli colleghi, dovesse essere considerata da noi retorica, lasciatemi dire che, allora, saremmo dei morti viventi, dei cadaveri in buona salute,

Si è tanto parlato in questi giorni di etica ed allora cerchiamo di inquadrare meglio come potrebbe essere il futuro e quale potrebbe essere la normativa che - si dice - verrà varata in tempi così brevi (ed io invidio coloro che in tempi così brevi riescono a trovare delle soluzioni).

la dottrina su cui si fondano i comportamenti del nostro agire, dell'agire comune. Ebbene, cambia il quadro di riferimento, deve cambiare anche il quadro etico generale. D'accordo, è un dovere morale del Parlamento ridefinire questi standard, è evidente a tutti che porre limiti in questa materia è oltremodo difficile. Faccio solo due riferimenti a due questioni specifiche. Il primo è il confine labile, assolutamente labile - checché se ne dica - tra eutanasia attiva e interruzione dell'accanimento terapeutico, cioè il lasciar morire serenamente. Il confine è estremamente labile. La seconda questione riguarda la differenza tra la sfera privata e la sfera pubblica entro cui accadono questi fatti drammatici. Ebbene, nella sfera privata abbiamo innumerevoli esempi di familiari, mariti, mogli che

di eutanasia attiva applicata proprio dai congiunti. In questo caso, ci si trova di fronte effettivamente ad un atto di eutanasia attiva, un atto di amore, per il quale poi si chiede il perdono della legge. è tutt'altra questione e attiene alla sfera privata. Trasferire questo concetto nella sfera pubblica è complicato e rischioso. È rischioso accettare per legge il concetto stesso di eutanasia attiva,

conoscete. A questa signora, proprio per una sentenza, è stata interrotta la respirazione artificiale. Gli esperti erano convinti che questo avrebbe comportato la rapida morte della signora, la quale invece ha vissuto per altri otto anni: semplicemente, gli esperti si erano sbagliati. Ma l'interruzione della respirazione era l'interruzione di una terapia, non era un atto irreversibile, tant'è che nessun nessun giudice ha emesso l'ulteriore sentenza di interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione. Questo è il punto, che secondo noi è fondamentale: lasciar morire, interrompere l'accanimento terapeutico, altra cosa è l'atto irreversibile dell'eutanasia attiva applicata mediante l'interruzione dell'alimentazione, che non ci trova assolutamente d'accordo.

vorrei dire al senatore Perduca che sarebbe il caso di approfondire bene il riferimento all'articolo 32 della Costituzione, che fa divieto delle cure sanitarie obbligatorie, ma sempre con riferimento al diritto fondamentale della tutela della salute. E questo è il passaggio principale che ogni tanto sfugge in merito a ciò che statuisce l'articolo 32. Può essere motivo di approfondimento delle sue riflessioni: niente cure obbligatorie per tutelare la salute, non per consentire il diritto di morire. È un concetto diverso, che la Costituzione comunque chiarisce bene nella prima parte dell'articolo 32.

Signor Presidente, vorrei innanzitutto premettere, nell'espressione del parere sulle mozioni, una considerazione, quella per la quale ciascuno di noi, qualunque posizione abbia avuto nel corso

e i modi con cui regolare la fine vita. Ho letto, in particolare, con attenzione la lunga e complessa mozione del devo fare un rilievo insieme positivo ed amaro: il combinato disposto delle mozioni dei due grandi Gruppi parlamentari di quest'Aula, se tradotto immediatamente in norme di legge, non consentirebbe più un caso Eluana Englaro. Nella mozione del Partito non soltanto si indica il dovere di fornire alimentazione ed idratazione fino all'ultimo momento di vita, ma proprio per questo non lo si considera terapia. Tuttavia, si prevede un'eccezione, quella cioè della possibilità di rinunciare all'alimentazione e all'idratazione attraverso una volontà espressa direttamente attraverso la dichiarazione anticipata di trattamento. Ciò a mio avviso costituisce una contraddizione in termini, ma comunque nega la possibilità di una rinuncia sulla base di una volontà presunta, volontà presunta, che è stata invece invocata dagli atti giudiziari che hanno consentito la conduzione a morte di Eluana Englaro. Quindi, la mozione del Democratico, nel momento in cui nega che possa trattarsi, nel caso di alimentazione e di idratazione, di trattamento nega il fondamento degli atti giudiziari in base ai quali è stata consentita la morte di Eluana Englaro. Troverebbe ragione, nelle mozioni che esprimono la grandissima parte di questa Assemblea, la considerazione che aveva condotto il Governo ad un provvedimento di necessità ed urgenza, quel provvedimento cioè che avevamo inteso adottare per impedire che Eluana Englaro fosse l'unica persona a morire sulla base di atti giudiziari, peraltro con le caratteristiche che sono state ricordate in quest'Aula da molti interventi, atti cioè di giurisdizione volontaria che, come tali, possono essere soggetti soggetti a cambiamento perché cambiano le condizioni di fatto e di diritto nell'ambito delle quali quei provvedimenti sono stati assunti. una considerazione positiva ma anche amara, perché il Parlamento, il Senato della Repubblica, che oggi si accinge ad esprimersi per la prima volta nel merito di questi temi, arriva tardi rispetto ad una persona che poteva e doveva essere salvata, rispetto ad un atto che la stampa internazionale oggi considera eutanasico, eutanasico, con tutta l'attenzione che merita questa novità - a mio avviso ovviamente tutt'altro che positiva - intervenuta nei comportamenti di questo Paese. Non posso, però, proprio per le ragioni che poco fa ho espresso, dare il parere favorevole del Governo alla mozione del Partito Democratico.

tuttavia, con un salto logico che mi permetto di sottolineare, nell'assoluto rispetto ovviamente per la posizione del Partito Democratico, riconosce la possibilità - attraverso dichiarazione espressa, certamente non presunta - di rinunciare rinunciare all'alimentazione e all'idratazione con una scelta anzitempo espressa seppure direttamente dalla stessa persona. Questo punto rimane un nodo che in sede legislativa dovrà essere sciolto e probabilmente costituisce il motivo di maggiore contrasto tra le diverse posizioni che si confronteranno nel corso dei lavori

certa e chiara che il Senato della Repubblica non potrà non riproporre nel momento in cui si esamineranno i testi legislativi che sono all'esame della Commissione igiene

che l'alimentazione e l'idratazione costituiscano un bisogno vitale e si afferma che esse rappresentano trattamenti medici. si impegna il Governo a proporre un provvedimento che, invece, opportunamente abbiamo rimesso al lavoro parlamentare. Auspico, quindi, un'espressione chiara della volontà dell'Aula, tale da incoraggiare un rapido percorso parlamentare per quanto riguarda finalmente la normazione della fine vita.

si conferma avere carattere di necessità ed urgenza anche all'indomani della morte della povera Eluana Englaro. Moltissime persone in Italia, potrebbero trovarsi ancora in quella stessa condizione, soggette ad analoghi provvedimenti giudiziari nel contesto di questo vuoto legislativo, e sono non soltanto le persone che si trovano in uno stato vegetativo persistente, ma anche le tantissime persone a loro assimilabili, come quelle affette

per le quali il Governo auspica provvedimenti utili a garantire una vita dignitosa, cui non può mai mancare l'alimentazione e l'idratazione.

un voto favorevole a nome del mio Gruppo su una vicenda in cui noi ci siamo mossi solo per il desiderio di mettere al primo posto la difesa della vita, comunque e sempre; un Gruppo che è amareggiato - come ha detto il nostro Presidente ieri - perché siamo giunti troppo tardi su un malato che non era un malato terminale e questo va sottolineato. Intervengo su un argomento - e questo forse è l'unico fatto positivo - che ha messo in evidenza in quest'Aula come molti di noi riconoscano più un'appartenenza a un fatto di coscienza, ad un orientamento intimo,

o è vita solo quando si ha un'autodeterminazione, una capacità di orientamento, o quanti tipi di vita esistono parallelamente. È vivo solo chi è capace di determinarsi, di muoversi, di fare quello che vuole e quindi non è vivo chi invece deve dipendere da altri, deve accettare l'aiuto di una suora misericordiosa, quando la trova? Alcuni colleghi hanno parlato di questa fascia intermedia, di cui nessuno può dire niente. niente. Alcuni dicevano che qualche neurologo sa tutto e probabilmente questo non è vero. Abbiamo visto che qualcuno ha rispolverato il limbo per collocare questo tipo di malati, che secondo lui non ha diritto a vivere, non è vivente. Noi, molto più umilmente, accettiamo l'ipotesi del saggio sindaco di Lecco, il quale sosteneva che questo è uno stadio di fragilità questo è uno stadio di fragilità e, in questi casi, non possiamo non essere lì vicino. La vita comunque va sempre difesa ed è vita comunque. consentite al collega di svolgere la sua dichiarazione di voto in un ambiente in cui possiamo tutti ascoltare. FOSSON Grazie, Presidente. Nessun medico, e qui ve ne sono molti, tra cui anch'io, può dire quale livello di coscienza e affettività era quello che viveva la povera Eluana.

La maggior parte dei medici, dei colleghi si è rifugiata in un dubbio, di fronte ad un argomento che non si può definire correttamente dal punto di vista scientifico. E il dubbio ha portato ad una norma precauzionale. Non sapendo che cosa era giusto o meglio fare, la precauzione era comunque salvare la vita, dare da mangiare e da bere a chi ne ne aveva bisogno, a chi non era un malato terminale, a chi non aveva una flebo e una terapia parenterale in atto. Lavoreremo sicuramente sulla legge sulla legge di fine vita, sul testamento biologico, mossi da questo desiderio comunque di salvaguardare la vita, riconoscendo e sottolineando la necessità di rispettare un ambito di libertà e di autodeterminazione,

l'occasione della dichiarazione di voto favorevole alla mozione di cui sono firmatario mi consente di esprimere pubblicamente una serie di riflessioni disordinate e anche emotivamente sofferte. Credo che questa esperienza ci abbia segnato tutti, soprattutto chi non aveva da rivendicare posizioni di parte per acquisire consenso politico, chi si è posto in questa vicenda con il rispetto che una storia così dolorosa merita, non soltanto per la povera Eluana, ma anche per una famiglia segnata da un dolore grandissimo,

troppe invasioni nella sfera personale, giudizi sui rapporti o sulle capacità affettive dei genitori: vi è una politica che invade il campo in modo assolutamente brutale. brutale. Questa vicenda così delicata, rispetto alla quale ognuno si pone con le ragioni finanche dei suoi princìpi religiosi, etici e morali, ha una sua complessità. E certo è opportuna la spinta che da essa viene per affrontare il tema di una disciplina attenta e prudente in questo campo,

assolutamente condivisibile, in cui anche e soprattutto la vicenda processuale, il modo in cui si è giunti all'esito, sollevava fortissime perplessità: la ricostruzione *ex post* in modo implicito di una volontà. Non so se debba essere annoverato tra gli ipocriti, ma anche la riflessione di Panebianco sulla sana ipocrisia, che consente di definire queste storie all'interno di una

Ambedue sollevano interrogativi ulteriori che vorrei comprendere come saranno sciolti anche nei lavori parlamentari. Se la volontà di Eluana non fosse stata ricostruita *ex post* in modo implicito ma fosse stata esplicita, sarebbe stato legittimo rinunciare all'idratazione e all'alimentazione forzata o il nostro ordinamento o il nostro ordinamento si appresta a considerare questo un obbligo che deve essere definito giuridicamente anche contro la volontà del soggetto? Ho sottoscritto la mozione e la voterò, perché la frase per quanto secca e dura che nessuno debba più morire di fame e di sete la condivido, sempre nella consapevolezza che non si riproduca un caso come questo, in cui una sentenza, un provvedimento giurisdizionale ricostruisca in modo implicito una volontà. Ma vorrei che su questa materia non si sviluppassero barriere ideologiche. Lo Stato che oggi viene chiamato a definire una disciplina sul testamento biologico, o meglio, sulla regolazione della fine vita deve essere uno Stato rispettoso, che sia a garanzia della persona, dell'individuo ed anche dei valori familiari e non uno Stato etico che debba imporre princìpi e valori con la certezza assoluta della verità. E lo Stato etico può essere una tentazione che alligna da ambedue le parti. E sono molto fiducioso che anche chi come me, in termini molto faticosi, fa riferimento e crede al messaggio cristiano trovi una Chiesa aperta, che ha definito in modo esemplare il principio dell'accanimento terapeutico evidenziando la necessità che l'onnipotenza tecnologica non degeneri in una una violazione della dignità dell'uomo. Considero l'accanimento terapeutico l'altra faccia dell'eutanasia, un'onnipotenza dell'uomo e della sua tecnologia che violenta la dignità della persona. persona. Questa vicenda drammatica pone interrogativi straordinariamente delicati a chi si vuole interrogare con onestà e con la consapevolezza della sua debolezza di uomo e non come assertore di princìpi assoluti

ma laicità non è laicismo, non è relativismo etico, non è abbandono dell'uomo: è rispetto dell'uomo. Ecco, credo che il percorso sia faticoso e che la drammaticità di questa vicenda ci debba consigliare prudenza, misura, rispetto e sensibilità. Dobbiamo tutti sfuggire agli eccessi di strumentalizzazione ed all'utilizzo di questa drammatica storia per perseguire altri obiettivi. Sarebbe il modo più serio di rispettare la memoria di questa giovane donna e il dolore, che io credo forte ed intenso, di una famiglia provata da un'esperienza, e che ha e che ha avuto forse il torto di volere che attorno a questa vicenda intervenissero le istituzioni. Come molti ci siamo infatti detti - non so se ipocritamente - che tutto sarebbe stato più semplice

cultura medica caritatevole. Ma, visto che il tema è stato posto alle istituzioni, esse devono rispondere con sensibilità, con intelligenza e con misura. Rimane confermato il mio voto favorevole alla mozione Gasparri, perché pone - e lo riconfermo - un caposaldo per quanto mi riguarda assoluto, e cioè che non debba più accadere che una persona venga privata di idratazione ed alimentazione senza il suo consenso.

quale ci ha richiamato stamattina perfino la Chiesa, perché dobbiamo far silenzio e dobbiamo pregare, nel rispetto e nella solidarietà verso la famiglia. Cercherò di affrontare invece i problemi di ordine generale che questo caso ci ha imposto. Devo però fare anche una premessa: credo che in questo dibattito ognuno di noi porti una storia personale, una propria cultura, un percorso;

convincimenti. Devo dire con estrema chiarezza che non ho apprezzato le gazzarre di ieri, né le accelerazioni imposte dal Presidente di questa Assemblea e dal Presidente del Consiglio su alcuni provvedimenti. Credo che questa compressione assoluta

Noi non vogliamo lo scontro istituzionale, lo abbiamo detto tutti. Per questo bisogna raccomandare ancora una volta di abbassare i toni,

spesso della Chiesa mi sembra un'altra di quelle vergognose strumentalizzazioni che non devono assolutamente essere fatte. Credo che il fariseismo e il doppiogiochismo, in questi due giorni, abbiano prevalso in quest'Aula,

alla mozione dell'Italia dei Valori addebitandole dei contenuti che non ci sono non sia una buona premessa. Dove sarebbe scritto che noi dichiariamo che l'idratazione e l'alimentazione sono terapie?

e dell'aborto. Non mi iscrivo tra quelle persone che dicono di essere contro l'aborto e poi praticano l'aborto clandestino, che dicono di essere

a cure pericolose o troppo onerose (...) che solo servirebbero a prolungare la vita in modo artificiale e penoso con danno del malato".

Esiste anche la morte naturale.

e, soprattutto, del rispetto per la morte. Avrebbe dovuto essere il giorno del silenzio ma, in realtà, siamo qui a rafforzare determinati concetti. Tutto dovrebbe essere fatto in assoluta serenità e senza polemica alcuna e questa è la mia intenzione. Non posso, però, non ripartire da alcune affermazioni fatte da alcuni colleghi che mi hanno preceduto, a partire dal senatore Pistorio, il cui intervento condivido appieno, e che va a ricollegarsi con l'intervento del senatore Perduca. Se Beppino Englaro avesse voluto decretare semplicemente la buona morte, l'accompagnamento con discrezione della figlia nell'aldilà, in questi anni avrebbe avuto più di mille occasioni per farlo privatamente, in ospedale, come normalmente avviene dappertutto: non dobbiamo scandalizzarci di questo. Evidentemente, è stata una scelta precisa, come ci ha detto espressamente il senatore Perduca, quella di trasformare un dramma privato in una crociata, giusta o sbagliata che sia,

ad avere perso in parte e in parte ad avere ancora una grande occasione. Io reputo che ieri sera abbiamo perso una grande occasione per sancire un principio *ex lege* da cui partire nelle disposizioni di fine vita. Abbiamo perso la possibilità di scrivere, definitivamente con una legge, che non sono assolutamente rinunciabili e sospendibili l'idratazione e l'alimentazione, per poi ripartire da lì per predisporre una legge globale, completa e che potesse dare un significato e una dignità alle disposizioni di fine vita. Non abbiamo avuto il coraggio di farlo. Ancora meglio, non tanto non tanto noi qui al Senato non abbiamo avuto il coraggio, quanto piuttosto una certa visone distorta - permettetemi di usare questo termine - della politica fuori da questa Aula ha fatto sì che questo processo si bloccasse. Non sto a giudicare ragionamenti politici di alto livello, che non mi competono e di cui prendo esclusivamente atto. Prendo atto del fatto che questa mattina, rispetto a ieri sera, facciamo venti passi indietro.

Si ricomincia però dal lavoro della Commissione e io vorrei esprimere l'esortazione a non farci prendere tutti quanti, in Commissione prima e nell'Aula poi, dalla smania della fretta

le disposizioni di fine vita che verranno emanate con questo provvedimento (non importa se ci vorrà una settimana o un mese di tempo in più) possano essere reali e non si debba mai più

non ci sono vincitori né vinti di fronte a un fatto di questo genere! La sconfitta è nostra, cioè del Parlamento, che si è lasciato prevaricare dalla magistratura, che come al solito non si limita ad applicare la legge tendenzialmente la interpreta e, questa volta, ha legiferato. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL)*. In *vacatio legis*, la magistratura ha legiferato passando sopra le nostre teste e la nostra volontà. Riprendiamoci il dovere ed il diritto di legiferare e promulgare una nuova legge.

è stato da tutti puntualizzato - non sono voluttuarie, non possono rappresentare scelte terapeutiche, perché sono di per se stesse un supporto irrinunciabile per la condizione minimale di vita di ogni individuo.

per quelli riportati ai numeri 8 e 11. Infatti, noi rifiutiamo l'obbligo di nominare un fiduciario, così come rifiutiamo la possibilità di introdurre nelle disposizioni anticipate di trattamento l'idratazione e l'alimentazione.

Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è venuto il tempo della responsabilità dopo il clamore di questi giorni, dopo il dolore e la morte. La compostezza della morte impone la compostezza ai vivi. È il tempo della responsabilità del Parlamento e i testi oggi al nostro esame ne sono espressione, impegnando il Senato a fare la sua parte, a colmare il grave ritardo, dando presto al Paese una legge che aiuti tutti a vivere con dignità e rispetto la fine della vita. La stessa dignità e lo stesso rispetto che si devono a ogni persona in ogni fase della vita. È il tempo della responsabilità del Parlamento, che vorremmo condivisa. L'avvio della discussione in Commissione e il dibattito pubblico ci consegnano una base di partenza buona per il confronto; tocca a noi ora arrivare ad un punto di sintesi, in un compito inedito nella storia democratica del nostro Paese, ma alla nostra portata se ci muoviamo nel solco della ragione, dell'umanità, dei valori che fondano la civiltà del nostro popolo, a condizione che si lavori con disinteresse fuori da ogni uso strumentale davvero non ammissibile. Su temi come questi, dove sono in gioco i passaggi e i valori ultimi dell'esistenza, con le sue speranze, i suoi smarrimenti e le sue paure, dentro le conquiste e le sfide della scienza e della tecnica, noi pensiamo che alla politica debba essere necessaria la virtù della misura, perché, come diceva Bonhoeffer, in tempi assai oscuri, quando viene meno il senso della qualità dell'uomo e la forza di mantenere le distanze, allora si è a un passo dal caos.

ne ha a lungo profondamente e appassionatamente discusso e la mozione oggi presentata ne costituisce l'esito, un primo esito. Una discussione che ha assunto il dialogo tra laici e cattolici chiedo scusa perché le parole non sono appropriate ma sono ancora quelle in uso - come un valore, come una opportunità storica per il nostro Paese, un elemento irrinunciabile nel solco dei valori costituzionali, di quella Carta costituzionale che promuove e difende le vita (senza questa Costituzione la vita sarebbe certamente meno tutelata), nel contesto delle pluralità e delle responsabilità in essa chiamate in causa: quella del cittadino nel suo diritto alla salute, alla scelta di fronte alle terapie; quella dei familiari; quella del personale medico e sanitario; quella di un Parlamento chiamato a interpretare una società pluralistica; quella dello Stato laico in cui l'autonomia della politica e la distinzione e l'equilibrio dei poteri sono l'unica vera garanzia perché siano effettivi il rispetto della dignità della persona, la tutela della vita, il bene comune. È la Costituzione il luogo dei valori e delle regole assunte con il patto degli italiani, e degli spazi riconosciuti ai soggetti: è il luogo dell'epifania dei valori condivisi nella storia del nostro Paese. La nostra mozione, come è stata bene illustrata, ha il suo fondamento nell'articolo 32, che considera, con il diritto alla salute, la personale assunzione di responsabilità del cittadino verso di sé nel momento della sua maggiore fragilità. Sembra una contraddizione ma non lo è, perché è lì che va riconosciuto il valore della sua volontà e non potrebbe essere altrimenti. È questo in fondo il senso delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario e insieme della loro non obbligatorietà, perché è anche nella libertà della persona un suo diverso affidamento al corso delle cose. Dichiarazioni anticipate di volontà in una cornice di garanzia, di appropriatezza, di praticabilità e di riconoscimento del principio di precauzione, i punti di arrivo di una lunga stagione della scienza e dell'etica. La nostra mozione ha il suo fondamento nel rispetto e nella tutela della dignità della fine della vita, nell'amorevole cura dell'intera società nei suoi confronti, anche sostenendo Colleghi, per cortesia, assumendo con il valore della vita anche il morire. Un piano che deve mettere queste cure a disposizione di tutti in ogni parte del nostro Paese. Qui c'è tutto lo spazio per l'impegno, anche finanziario, del Governo. Ha il suo fondamento la nostra mozione nel riconoscimento della libertà della coscienza e dell'obiezione di coscienza, che ne è parte. Ha il suo fondamento nell'esclusione di una qualunque forma di eutanasia, di accanimento terapeutico, di abbandono terapeutico. Noi vogliamo trasformare la nostra società perché diventi una società alleata della vita, a partire dall'alleanza terapeutica medico-paziente. Alziamo lo sguardo: l'Italia ha bisogno di fiducia, di impegno condiviso, di pace religiosa. Ma il punto di partenza è il rispetto degli uni verso gli altri e di tutti verso le persone, soprattutto verso coloro che soffrono. Quando sono così palpabili i sentimenti più profondi, quando siamo di fronte alla vita che incontra in modo così ravvicinato il suo limite, la morte, e lo comprende, è più forte il diritto alla dignità e alla pace della morte. Di assoluto nella vita degli uomini vi è soltanto l'amore, come Antigone ci insegna. Anche una buona legge può essere un contributo, e un contributo importante, ma senza ambizioni di onnipotenza né per la legge né per la scienza né per la tecnica. Qui siamo legislatori avendo presente, come dice la Carta, la dimensione universale del valore della persona e del bene comune. Siamo qui impegnati con tutto noi stessi, con la nostra vita, con i nostri valori, con la nostra storia. Siamo impegnati con la nostra coscienza, che su questi temi è la prima, direi l'unica cifra della politica. A cominciare dal Partito Democratico con piena e pari legittimità per tutte le opinioni; una coscienza libera di fronte alle scelte, anche politiche, e responsabile, che comprende anche la scelta, il tentativo di cercare insieme, comunitariamente, la costruzione di obiettivi condivisi. Questo è il grande valore della politica: dentro il Partito Democratico, in quest'Aula e nel Paese. La libertà di coscienza individuale comprende sempre anche questo sforzo, al di là dei risultati. La mia coscienza, colleghi, si è formata nell'Italia democratica e nella Chiesa del Concilio; con gioia, senza contraddizione e con gratitudine per entrambe. A molti, a molte, laici e cattolici, sono grata per avermi formato ad assumere responsabilità e ad assumerla soprattutto nei momenti difficili, non scontati. Quanto è grande, colleghi, il cammino della storia; molto più grande di noi, ma senza di noi non avanza. Quanto si carica sulle nostre spalle la responsabilità dei passi che aprono il nuovo cammino che l'Italia attende. Abbiamo fiducia, colleghi. Penso che possiamo essere all'altezza del compito. Abbiamo il dovere di esserlo. Può partire di qui un passo nuovo per la politica italiana, per la sua efficacia, per la sua credibilità, per l'innalzamento del suo livello di confronto. Il nostro è un tempo assai difficile, ma è il tempo nostro. Per me, lasciatemelo dire, è anche un tempo di grazia.

Signor Presidente, è davvero difficile per me intervenire dopo un intervento così vero e vibrato,

avrei preferito un testo migliore. Preferirei che quel di troppo di provocazione che è nell'ultima riga e mezza della premessa venisse tolto, ma tant'é, in quel dispositivo c'è il mio pensiero, c'era il mio pensiero ieri, c'è il mio pensiero oggi e ci sarà il mio pensiero domani. Non mi appartiene e trovo ostica questa distinzione tra politico, credente, cattolico, laico. A me tocca la fatica quotidiana di una sintesi tra ciò in cui credo e ciò che devo fare. Non so se sono in perfetta solitudine, questa mattina, ma quella sintesi mi dice di volta in volta qualche volta in maniera felice, qualche volta meno - qual è la parte che devo fare e la parte che mi sento di fare questa mattina è questa. *(PD)*. Signor Presidente, intervengo anche a nome della senatrice Poretti. Ringrazio la senatrice Soliani, che ancora una volta è riuscita a nobilitare le parti finali del nostro dibattito, e annuncio la nostra astensione con la non partecipazione al voto Il senatore Rizzi ha chiaramente messo a verbale che in questo Paese esiste l'eutanasia: dire no all'eutanasia non vuol dire cancellare il fenomeno. Non siamo mai stati a favore del divorzio, né dell'aborto, né dell'eutanasia; siamo a favore dell'adozione di una legge che consenta il governo e la regolamentazione di questi fenomeni, di modo da applicare la Costituzione garantendo il diritto di libertà. Non parteciperemo quindi al voto quando verrà messa in votazione la mozione del Partito Democratico. Voteremo invece contro tutte le altre.

le mie espressioni di dissenso di ieri pomeriggio rispetto al solo punto cruciale che trova largamente il Partito Democratico concentrato sulla difesa e sulla valorizzazione del primato della coscienza e della libertà individuale, a me pare che vi sia una insormontabile preoccupazione di consegnare alimentazione e idratazione alla sfera della obbligatorietà del sostegno vitale. Purdistinguendomi nettamente dalla modalità e dalla dalla concezione che anima molta parte della discussione e della indicazione pratica sottostante alla mozione presentata

Non è l'unico articolo della Costituzione pertinente per decidere la questione che abbiamo al nostro esame, e anzi sono un po' colpito che altri articoli non siano stati ricordati, ma è certamente un articolo rilevante.

esiste una libertà terapeutica di scegliere o di rifiutare le cure. Recita l'articolo 32: «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario». secondo punto è che l'articolo 32 afferma che questa libertà terapeutica, di scegliere o non scegliere cure, può essere vincolata da una legge: «Nessuno può può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». È evidente perciò che una legge può consentire l'esercizio positivo della libertà di cura o di rifiuto della cura. è poi un terzo punto nell'articolo 32 che è importante quanto gli altri due: qualunque legge si voglia o si debba fare in ossequio all'articolo 32, qualunque legge sulla libertà di curarsi o sul rifiuto delle terapie, qualunque legge ha un limite; e la nostra Costituzione dà un nome, ripetutamente, a questo limite. L'articolo 32 chiama questo limite rispetto della persona umana; l'articolo 41 della Costituzione introduce un'altra espressione equipollente per nominarlo e parla di dignità umana; e poi c'è l'articolo 2,

per ricordarlo in primo luogo a me stesso, dice, dando il nome a quel limite invocato anche dall'articolo 32: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo». Sono espressioni molto serie, sono espressioni molto gravi. «Riconosce e garantisce» significa che la Repubblica non li crea questi diritti inviolabili dell'uomo,

sono diritti che esistono prima dell'esistenza di una comunità politica o statale, sono diritti che stanno lì e che la Costituzione, il Parlamento, la comunità politica, deve solo riconoscere, cioè prenderne atto, dai Gruppi PdL e LNP).* E sono inviolabili, cioè non negoziabili, non cedibili, non modificabili: sono diritti assoluti, preesistenti, legati all'uomo in quanto uomo. Ecco il nome proprio del limite fissato dall'articolo 32 della Costituzione. Ora, la questione che qui si pone e che è stata dibattuta in questi giorni, in queste ore, e per tanto tempo anche, è se violare la vita di una persona, consentire ad una persona in stato terminale di porre termine ai suoi giorni, sia o no una violazione dei limiti posti dagli articoli 32 e 2 della Costituzione.

anche il diritto alla vita è disponibile quando la vita non è più vita e non ha più dignità di vita. Io credo che qui vi sbagliate: credo che dicendo così vi poniate fuori dall'articolo 32 e dall'articolo 2, perché quel paziente terminale, quel paziente in coma permanente, quel paziente che non ha più scientifiche e ragionevoli speranze di vita, quel paziente è ancora un uomo che ha la sua dignità

esprimiamo sofferenze. Quel paziente è un individuo che chiede la nostra comprensione, la nostra solidarietà, la nostra pietà, che instaura con noi una comunità. Perciò è un uomo che, in quanto uomo, per l'articolo 2 della Costituzione italiana ha diritti inderogabili, inviolabili, noi non possiamo toccare. Quei diritti non sono violabili e non li può violare né il paziente medesimo in qualunque momento della sua esistenza, né i suoi genitori, né la magistratura, né il Parlamento; sono, appunto, inviolabili.

Voi usate anche un altro argomento a cui ho prestato molta attenzione; voi dite che in realtà lasciar morire, e perciò violare, sia pure eccezionalmente, il diritto fondamentale di quell'individuo, in realtà è consentito perché così facendo si rende un tributo alla sua libertà individuale. È un argomento che ha svolto in quest'Aula in particolare il senatore Veronesi: la libertà individuale. Ho ascoltato l'intervento del senatore Bosone, che era palesemente in replica e di critica a quello del senatore Veronesi, e dico che vi sbagliate anche su questo punto. Togliere l'alimentazione ad un paziente, sia pure quando quel paziente non ha più ragionevoli speranze di vita, significa togliere la vita e togliere la vita significa togliere il presupposto della dignità; ma se significa togliere la dignità, allora lì c'è la violazione di un diritto che è inalienabile. Mi chiedo poi quale concetto è mai quello che viene introdotto di libertà individuale. Cos'è questa libertà individuale che è garantita entro certi limiti dall'articolo 32? La libertà individuale vuol dire forse discrezionalità assoluta? discrezionalità assoluta? La libertà individuale vuol dire arbitrio? La libertà individuale vuol dire licenza di fare di sé e degli altri ciò che si crede o la libertà individuale è sempre accompagnata dalla responsabilità? Confondere la libertà individuale con l'arbitrio, con la licenza significa passare dalla civiltà della ragione alla barbarie dell'egoismo.

nell'articolo 2, nell'articolo 32 e nell'articolo 41 della nostra Costituzione per dire che non possiamo sottrarre l'alimentazione a chi sta per lasciarci.

Non ho nemmeno introdotto alcun riferimento alla Chiesa cattolica,

argomenti. Per i laici autentici, per quanto riguarda la religione, basta la religione dell'articolo 2 della Costituzione; è sufficiente per prendere le nostre decisioni. È la religione di quell'articolo 2 che stabilisce che siamo tutti uguali in dignità, abbiamo tutti gli stessi diritti fondamentali rispetto a quella dignità. C'è stato un tempo, cari amici, che i laici non avevano timore di dare un nome alla religione dell'articolo 2 della Costituzione; avevano il coraggio di darlo, quel nome. La religione dell'articolo 2 della Costituzione è la religione cristiana. Oggi molti laici lo hanno dimenticato, oggi molti laici credono che questa religione sia di ostacolo, credono che l'interprete di questa religione, cioè la Chiesa cattolica, sia di impedimento o interferisca, credono che senza quella religione noi saremmo più liberi, renderemmo più omaggio alla libertà individuale. È un altro grave errore. I laici hanno bisogno, per decidere su argomenti come questi, della religione dell'articolo 2. Sanno da dove viene quella religione dell'articolo 2, ne sono fieri, sono disposti a testimoniarla e a difenderla. Altri laici, invece, affievoliscono la consapevolezza della religione dell'articolo 2 (il senatore Ichino parlava di una generica tradizione biblica), oppure ritengono la religione cristiana un ostacolo. Noi la pensiamo diversamente, non abbiamo bisogno di nessun ammaestramento, di nessun magistero: la Costituzione ci dà i parametri giuridici e culturali sufficienti per prendere le nostre decisioni. Chi volesse decidere diversamente

che è bene non sospendere l'alimentazione e l'idratazione sia il modo concreto per esprimere un sì convinto alla vita,

Non condivido inoltre la mozione della maggioranza, perché, per quanto l'abbia letta e riletta, non dice nulla.

non potrò neanche votare la mozione del Partito Democratico in quanto non condivido una parte essenziale del punto 11) della mozione stessa. Per il motivo precedentemente apre una nuova finestra"). Prima di passare alla votazione, avverto gli onorevoli colleghi che le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni. Passiamo quindi alla votazione della mozione n. 86

che garantiscano la certezza di cure idonee e di adeguata assistenza nella fase terminale dell'esistenza ovvero quando le condizioni personali non consentano di provvedere in maniera autonoma alle necessità vitali fondamentali,

legislativa in materia di fine vita, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possano in alcun caso essere negate da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

che è preclusa nella parte del punto 11) che recita: «nonché la previsione che nell'ambito del principio di autodeterminazione è ammessa l'eccezionalità dei casi in cui la sospensione di nutrizione e idratazione sia espressamente oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento; 12) la promozione di campagne

sospendere la nutrizione e l'idratazione nel caso di volontà espressamente dichiarata anticipatamente. Permangono tuttavia per il Governo ragioni che lo portano ad esprimere un parere contrario, tra le quali rilevo mozione, laddove si prevede la "nomina obbligatoria di un fiduciario o curatore che agisca nell'esclusivo interesse della persona che gli ha dato mandato attuandone la volontà espressa nella dichiarazione Ci sono poi anche altri elementi, certamente meno rilevanti del punto che è stato, come abbiamo detto, definito poco fa dall'Aula. Per tali motivazioni, ribadisco il parere contrario

Per cortesia. Prego, senatore Bricolo, continui il suo intervento. BRICOLO *(LNP)*. «Famiglia Cristiana» scrive in questo articolo che siamo alle leggi razziali.

ma visto che il Parlamento è stato chiamato a votare una legge sull'immigrazione, un tema difficile che ci ha visto confrontare in Commissione per diversi mesi, credo che nessuno possa permettersi di attaccare l'istituzione Senato, perché in questo Paese non si fanno leggi razziali. Le norme che abbiamo emanato e che sono contenute in quel disegno di legge sono norme già applicate nella stragrande maggioranza dei Paesi europei.

declinare in maniera diversa. Voglio condannare recisamente il metodo con il quale i Gruppi di maggioranza, fino a pochi minuti fa, si sono preoccupati di spiegare a noi dell'opposizione come fossimo sottilmente e sostanzialmente distanti e contrari rispetto alle posizioni della Chiesa e poi, rispetto ad una legittima critica che proviene dal mondo cattolico e da un suo giornale tradizionalmente austero e importante, si arrivi, da parte degli stessi colleghi della maggioranza,

ragione sono contrario a qualsiasi intervento di carattere censorio, anche quando si utilizzano toni che non sono quelli che per cultura appartengono a ciascuno di noi e quando sono eccessivi, ma mi piacerebbe che si utilizzasse lo stesso metro e la stessa misura per tutti. conclusione, credo che sia stato introdotto in quest'Aula in maniera irrituale un dibattito su una critica, ancorché legittima, ad una via che «Famiglia Cristiana» ha usato per manifestare la sua opinione, un'opinione che nel contenuto noi condividiamo.

più caute, prudenti e rispettose anche quando dobbiamo far valere legittimamente opinioni diverse. da «Famiglia Cristiana» è delicato. Questo ramo del Parlamento ha legiferato, e io ho votato quelle norme, tuttavia accetto le critiche di tanta parte, non solo del mondo cattolico, ma anche del mondo medico, perché è una materia delicata in cui il legislatore ha compiuto una scelta, che non ci esime dal diritto di critica di altri. Io credo, rispetto alla Chiesa cattolica che tanto spesso viene invocata in modo quasi militante, che sia necessario accettare la complessità e la ricchezza di quel mondo, in cui non vi è una voce univoca tranne quando si esprime il magistero papale. papale. Un rapporto corretto con il mondo cattolico è un rapporto dialettico e reciprocamente rispettoso. Questo è quanto intendo suggerire ai miei colleghi.

tutti dovremmo abbassare i toni, perché non si può mettere in discussione la libertà di stampa, anche quando è riferita a notizie che non ci fanno comodo.

Mi sembra che l'opinione espressa in una rivista sull'operato del Parlamento sia, appunto, un'opinione politica cui si può politicamente replicare. Su tale questione,

che ormai è una consuetudine parlamentare. È un decreto che di solito è semestrale (ve ne è, cioè, uno per ogni semestre) che provvede, appunto a prorogare alcuni termini con diverse motivazioni. È evidente che sarebbe preferibile, come sempre, un intervento anticipato che non rendesse necessaria una decretazione su questo argomento. Sappiamo bene, però, che, data

davvero una necessità generata dalla grande massa di norme che ci si trova non soltanto ad avere in vigore ma ad avere anche in via transitoria (perché stanno perdendo perdendo la loro vigenza o perché stanno entrando in vigore). In questo ambito, il Governo ha presentato una serie di provvedimenti, motivati da varie necessità: alcuni sono motivati anche dalla necessità di studiare meglio delle norme per poterle far entrare in vigore nel momento in cui siano state migliorate e rese più rispondenti alla realtà dei fatti. In Commissione, partendo da questa premessa (la quale implica anche il fatto che all'interno di questo provvedimento ci siano norme riguardanti materie davvero molto varie; ed è apprezzabile, sotto questo punto di vista, che

altre norme sotto forma di articoli aggiuntivi. È stato un lavoro positivo che ha richiesto

mantenere il controllo della spesa pubblica in una situazione di crisi internazionale, dove la nostra credibilità deriva, tra le sue fonti principali, proprio dalla capacità della pubblica amministrazione, del Governo, del Parlamento e degli enti locali di saper tenere sotto controllo la spesa. Da ciò dipende la credibilità dei titoli del debito pubblico e, di conseguenza, il tasso che lo Stato deve pagare su questo stesso debito, che sappiamo essere molto ingente per un'eredità dei decenni passati. Su tale binario è andata avanti la Commissione. Io confido che il lavoro svolto in quella sede sia recepito

che riguardano, ad esempio, le energie rinnovabili, in particolare da biomassa, che riguardano l'attività sia artigianale sia industriale ma anche agricola.

le comunicazioni che devono essere effettuate per quanto riguarda i rapporti di lavoro di carattere stagionale, anche su questo credo si possa e si debba intervenire per far fronte a picchi imprevisti di attività, specialmente nelle aree turistiche - penso alla mia area di montagna, ma anche alle aree lacustri

Presidente, prima di entrare nel merito specifico del provvedimento, come si presentava all'inizio e come è stato modificato dalla Commissione,

e si è compresso in qualche modo il diritto di iniziativa dei singoli parlamentari, perché si è posta in essere una legislazione concentrata sui decreti; il risultato di questa operazione è paradossale, nel senso che per bilanciamento vengono rigonfiati, crescendo a dismisura,

associativa sovracomunale; 5.2, che fa retroagire al 1999 anziché al 2001 la validità delle graduatorie concorsuali per i concorsi svolti dalle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni; a limitazioni delle assunzioni; 20.0.1, che proroga di ulteriori venti mesi i termini previsti per la cessazione di talune attività svolte nei confronti di soggetti pubblici da società partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali;

relativo alla proroga, fino al 2010, dei termini per la regolarizzazione catastale dei fabbricati rurali. Questa è la prima parte del ragionamento: gli emendamenti del Gruppo PD che sono stati approvati in Commissione. del Partito Democratico ha contribuito insieme alla maggioranza a due altri emendamenti molto positivi. Con l'emendamento 21.0.22 ci si è prefissi di evitare le conseguenze negative

di soprassedere ad ulteriori interventi su materie eterogenee, inadatte ad essere ricomprese nel decreto e/o con effetti comunque negativi, tra cui ne cito tre: la posticipazione del riordino degli enti di ricerca; la rinuncia a riformare la giustizia amministrativa e il relativo consiglio di presidenza; la rinuncia a un intervento sbagliato ed elettoralistico sulla Regione Sardegna. In quarto luogo, restano ancora per l'Aula da affrontare alcuni limiti rilevanti, tra i quali quelli più importanti, oggetto dell'iniziativa emendativa del Partito Democratico, non modificati dal testo originario, che sono

22.1, concernente il ripristino della norma interpretativa con la quale si consente la chiusura del contenzioso previdenziale dei datori di lavoro del settore agricolo operanti nelle zone di montagna e nelle aree svantaggiate; 22.0.1, che contiene la proroga delle agevolazioni contributive per il settore agricolo in aree svantaggiate e località montane; 24.1, che propone la soppressione, per ragioni di sicurezza, della proroga dell'entrata in vigore delle norme sulla limitazione alla guida per i neopatentati; 32.2, recante la soppressione della proroga dell'entrata in vigore di talune norme della legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 35.2, che propone l'estensione delle misure di stabilizzazione del personale precario oltre l'ambito degli enti di ricerca; 37.0.400, che propone la proroga della validità dell'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti dal Ministero dell'istruzione; 41.400, recante la soppressione della proroga, anche per gli anni successivi al 2008, del divieto per le pubbliche amministrazioni di estensione del giudicato; volto ad ottenere la soppressione dei nuovi poteri attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di bilancio dello Stato; 43.0.420, che propone il riconoscimento di trattamenti speciali di disoccupazione per i lavoratori frontalieri

In quinto luogo, sono da modificare alcuni emendamenti peggiorativi introdotti in Commissione. In particolare, si tratta degli emendamenti: 21.0.17, che rischia di peggiorare la qualità del servizio elettrico per i clienti delle imprese con meno di 5.000 utenti; 5.000 utenti; 29.0.1, che introduce modifiche in materia di concessioni autostradali del tutto estranee all'oggetto del provvedimento e che dovrebbero essere oggetto di accurato approfondimento nella Commissione di merito, cioè l'8a; 29.0.2 e 29.0.3, che prorogano l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di tecniche per le costruzioni e l'obbligo di installazione di impianti energetici solari nelle nuove costruzioni;

35.0.11, che introduce nuove modalità di accertamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito; 37.0.2, che modifica i meccanismi vigenti per la valorizzazione del percorso scolastico per l'accesso ai corsi universitari; 44.0.3 del Governo, relativo all'edilizia carceraria, che sposta risorse dalla Cassa delle ammende, finalizzata al reinserimento dei detenuti, per contribuire al pur giusto obiettivo di realizzare nuove carceri. Infinedevo dire che, superato

abbassando il livello di tensione ideologica, cosa di cui penso abbiamo tutti bisogno. Signora Presidente, intervengo in discussione generale anche per ottimizzare al massimo i tempi di lavoro di quest'Assemblea, dedicando questo tempo, che verrà risparmiato successivamente, all'illustrazione

Per questo motivo, mi rivolgo al relatore, e soprattutto al sottosegretario Giorgetti, per caldeggiare nuovamente la possibilità che questo emendamento venga accolto. L'emendamento 35.0.7

doveva servire per il pagamento di eventuali ammortizzatori sociali, soprattutto le casse integrazioni, dei lavoratori italiani in Svizzera, i frontalieri, che vengano a trovarsi nelle condizioni di perdita del proprio posto di lavoro.

Il grosso rischio è che questo fondo, che è stato alimentato, ripeto, dai frontalieri con versamenti provenienti dal proprio stipendio, venga utilizzato per altri scopi; e non potrebbe essere che così,

del *referendum* che sancisce definitivamente la sottoscrizione dei cosiddetti patti bilaterali tra Svizzera e Comunità europea, e il successivo recepimento, sempre da parte della Confederazione elvetica, di alcune normative europee per quanto riguarda la circolazione delle forze lavoro.

per far sì che vi fosse da parte dello Stato italiano una copertura per questi cittadini italiani lavoranti all'estero) ma dal 1° giugno 2009 alla cassa integrazione e agli altri ammortizzatori sociali per i frontalieri dovrà provvedere,

a favore di un particolare gruppo di lavoratori frontalieri che sono andati in pensione dopo l'anno 2000, subendo con ciò un'ulteriore beffa determinata dall'impossibilità

l'altra metà dei fondi (che, ripeto, non potrebbero mai più essere utilizzati dall'INPS o dal Tesoro per il pagamento della cassa integrazione: non ve ne sarebbe più la necessità, in quanto dovrà farsene carico la Confederazione elvetica),

scritto, per iniziative non solo culturali e sociali ma anche infrastrutturali che vadano a beneficio del frontalierato. Ovviamente non ne beneficeranno direttamente coloro che hanno versato i contributi al fondo ma sicuramente tutti i frontalieri che, ripeto, sono 42.000.